L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta

Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo preliminarmente di evidenziare come il CETA, l'accordo economico e commerciale globale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri da un lato e il Canada dall'altro, prevede sia la registrazione e la protezione di indicazioni geografiche originarie degli Stati membri dell'Unione europea in Canada - fra le quali quelle italiane - sia la possibilità di aumentare in futuro il numero delle indicazioni geografiche protette in Canada. In relazione all'asserzione dell'interrogante circa l'inefficacia dell'accordo contro la contraffazione alimentare, evidenzio che la tutela della qualità e della certificazione dei nostri prodotti di eccellenza esportati sul mercato canadese è assicurato dalla protezione che, ai sensi del CETA stesso, è stata garantita alle indicazioni geografiche inserite in un'apposita lista allegata al medesimo. Con tale disposizione il Canada, tradizionalmente estraneo a questo tipo di sistemi in quanto orientato al sistema dei marchi, ha riconosciuto un certo numero di indicazioni geografiche europee, di cui 41 italiane che, peraltro, rappresentano circa il 90 per cento del valore delle nostre esportazioni DOP e IGP in Canada e si aggiungono a quelle dei vini, già riconosciute e protette. Trattandosi peraltro di lista aperta, come più sopra accennato, quest'ultima potrà essere integrata successivamente con nuove indicazioni geografiche che dovessero essere riconosciute a livello europeo tramite una decisione assunta dal Comitato previsto dal CETA. Ulteriormente il Canada, a seguito della modifica della propria legge sui marchi, ha previsto la possibilità di ottenere una tutela anche per le indicazioni geografiche già esistenti in Unione europea, ma non presenti nell'allegato all'Accordo, previa richiesta diretta al Canadian intellectual property office. Sin dal primo giorno di applicazione provvisoria del CETA, pertanto, le 125 indicazioni geografiche europee hanno cominciato a beneficiare di una piena tutela attraverso l'Accordo e tale risultato ha permesso di risolvere il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione di alcuni dei nostri prodotti di eccellenza agroalimentare. Quanto alle indicazioni geografiche per le quali è stata prevista la coesistenza con marchi già registrati precedentemente in Canada (in particolare, Parmigiano Reggiano, tre prosciutti italiani e tre nostri formaggi), questa soluzione, individuata per tutelare i diritti acquisiti dagli operatori locali, ha comunque consentito la protezione di alcuni prodotti europei considerati fino ad allora «nomi generici», oltre a permettere la commercializzazione di alcuni prodotti, in particolare il prosciutto di Parma. Quest'ultimo, infatti, prima del CETA non poteva essere immesso sul mercato canadese con il suo nome, ma solo come «*original* prosciutto», data l'esistenza di un marchio «Parma» registrato quarant'anni prima. Inoltre, l'Accordo contiene specifiche disposizioni contro l'*italian sounding*, quali il divieto di evocazione per i prodotti non originari (ossia il divieto di uso di simboli, foto, colori e simili che possano evocare l'origine dell'indicazione geografica), l'obbligo di indicare l'origine sull'etichetta in modo chiaro e visibile, l'obbligo di ulteriore differenziazione per i prodotti introdotti sul mercato dopo una certa data, che dovranno riportare la dicitura «*style/imitation*» e così la possibilità di ricorso amministrativo da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale delle singole indicazioni geografiche. Per quanto sopra premesso, dunque, e con riferimento all'ulteriore rilievo dell'interrogante in merito al momento di importazioni nell'Unione europea di prodotti a denominazione «Parmesan» di origine canadese, si evidenzia come la legislazione europea ne vieti espressamente la commercializzazione, in quanto il termine «Parmesan» non è generico, ma rappresenta un'evocazione della denominazione «Parmigiano Reggiano» e come tale non può essere utilizzato in Unione europea per formaggi non conformi al disciplinare della DOP italiana. Eventuali casi di importazione di importazione che violino il diritto esclusivo nell'Unione della DOP «Parmigiano Reggiano» e dei suoi sinonimi possono essere segnalati alle competenti autorità degli Stati membri - nel caso dell'Italia, è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero ai sensi del regolamento unionale n. 1151/2012 - che hanno l'obbligo di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle Indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate nello Stato membro. Disposizione questa che è stata fortemente voluta proprio dall'Italia in quanto finalizzata a responsabilizzare le autorità degli Stati membri. Peraltro, il regolamento UE n. 608/2103 assicura la protezione doganale di tutti i diritti di proprietà intellettuale - incluse le indicazioni geografiche - registrati nell'Unione europea. Ma anche lo stesso Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano - è necessario evidenziarlo - svolge, come tutti i consorzi riconosciuti ai sensi di legge, una costante azione di controllo nel mercato unico, legittimata anche dall'articolo 54 del citato regolamento UE n. 1151/2012, segnalando casi di violazione del diritto, direttamente o mediante l'ICQRF, alle autorità competenti degli altri Stati membri. In relazione poi alla tematica della tutela dei prodotti sul mercato italiano e del rispetto dei requisiti di etichettatura a tutela del consumatore, faccio presente che l'offerta di informazioni chiare, comprensibili e leggibili sugli alimenti a tutela dei consumatori - materia armonizzata a livello europeo, dove il regolamento UE 1169/2011 assicura un elevato livello di protezione del consumatore, disciplinando tutti gli aspetti riguardanti l'etichettatura - è argomento di massima rilevanza e impegno per questo Ministero. Ne è riprova, ad esempio, la lettera sottoscritta a marzo scorso congiuntamente dal ministro Bellanova e dal Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, inviata ai commissari europei alla salute e all'agricoltura, in cui l'Italia chiedeva che venisse esteso l'obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, a partire da una scelta rapida sui prodotti sui quali si è già sperimentato in questi anni come latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso, derivati del pomodoro. In quest'ottica i suddetti Ministri hanno notificato a Bruxelles la proroga fino al 31 dicembre 2021 del decreto 9 dicembre 2016 su latte e formaggi e hanno poi firmato il decreto ministeriale del 1° aprile 2020, che proroga anche le disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro al 31 dicembre 2021. Ciò nella convinzione che nella strategia Farm to fork l'origine obbligatoria debba essere un tema centrale, proprio perché visto che quella locuzione si traduce «dal campo alla tavola», l'origine obbligatoria declina al meglio questa esigenza, affinché in etichetta il consumatore abbia la percezione dell'intero percorso di tracciabilità. Quanto poi alle attività di controllo, con riferimento specifico a quella posta in essere dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quest'ultima è improntata alla massima attenzione nella verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari. Ciò anche con controlli a campione di rintracciabilità, per accertarne la veridicità, contrastare il fenomeno dell'*italian sounding,* per tutelare il *made in Italy* e le produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell'Unione europea (prodotti DOP e IGP). Tramite i sistemi di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri Administrative assistance and cooperation system (AAC) e Food fraud network (FF), di cui I'ICQRF è punto di contatto per l'Italia insieme al Ministero della salute, vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri concernenti le irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura. Anche sul commercio via *web* a livello sono stati siglati specifici protocolli d'intesa con le principali piattaforme commerciali *on line* (eBay, Amazon, Alibaba), rafforzando la tutela dei consumatori che si avvalgono delle suddette piattaforme *e-commerce*, nonché la promozione, la valorizzazione e l'informazione sulle produzioni italiane DOP affinché nel mercato *on line* siano contrastati i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane di qualità. A fronte poi delle perplessità manifestate dall'interrogante in merito al fatto che la ratifica del CETA da parte dell'Italia - invece di rappresentare un'opportunità per la nostra Nazione - si concretizzerebbe, al contrario, in un veicolo facilitatore dell'importazione di prodotti agroalimentari con *standard* di sicurezza inferiori a quelli europei, rispondo evidenziando che tutti i prodotti agroalimentari provenienti dal Canada dovranno ottemperare alle normative europee in materia sanitaria e fitosanitaria, ivi comprese le norme che regolamentano l'accesso di organismi e prodotti geneticamente modificati. Analogamente, in ragione del principio di precauzione - che, previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 191, è obbligatorio e non può essere modificato o abrogato da alcun accordo internazionale, incluso il CETA e delle normative sanitarie e fitosanitarie, i prodotti trattati con sostanze vietate in quanto nocive (ad oggi, l'uso del glifosato è ancora autorizzato nell'Unione europea) o di cui non si ha evidenza scientifica sulla nocività, ma di cui si sospetta qualche rischio per la salute umana, non potranno accedere al mercato interno dell'Unione europea. Pertanto, posto che resta valido quanto già detto sul principio di precauzione, l'Unione europea continuerà ad applicare la sua legislazione sul divieto degli ormoni per allevamento animale, secondo quanto previsto dalla direttiva In aggiunta, l'importazione di carne non trattata da Paesi terzi che utilizzano per il loro mercato interno ormoni per allevamento è possibile solo nel caso in cui sia assicurata la segregazione degli allevamenti, principio che si applica anche all'uso degli antibiotici vietati nell'Unione europea, come previsto dalla direttiva 96/23/EC. Il CETA non ha ovviamente modificato il quadro normativo. Questo principio è stato per chiarezza riaffermato nelle dichiarazioni allegate alla procedura del Consiglio europeo per l'adozione della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell'Unione. In ultimo, per quanto, invece, attiene specificatamente alla tematica degli OGM, è opportuno ricordare che, con l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, è stato sancito il definitivo divieto di coltivazione di tutte le varietà di mais MON810 in Italia (decisione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016) e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio. La coltivazione di suddetti mais transgenici, autorizzati o in corso di autorizzazione, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 224. Ad oggi, non è stata presentata alcuna nuova richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per la coltivazione di nuovi OGM, né per il mais, né per altre specie. Pertanto, l'attuale sistema legislativo consente di intervenire su tutti i nuovi OGM per i quali viene chiesta l'autorizzazione europea alla coltivazione e al contempo il sistema sanzionatorio è in grado di punire tutti i possibili casi di violazione delle norme in vigore. Per quanto concerne la normativa sui sistemi di etichettatura degli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati, si ricorda che i prodotti, siano essi alimenti o mangimi, costituiti, contenenti o derivati da OGM, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003. Ciò garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole. Con il regolamento (CE) n. 1829/2003 viene stabilito che gli alimenti derivati da OGM, destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM. Inoltre, con il regolamento n. 1830 del 2003 gli alimenti geneticamente modificati devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità, definita come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dall'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

prima di entrare nel merito dell'interrogazione, molto interessante, è doveroso sottolineare

più simpatica è che giunge nel momento in cui non c'è più il Ministro delle politiche agricole. Come lei sa, da ieri non è più Ministro della Repubblica e probabilmente, tra qualche ora, non ci sarà nemmeno più un Governo che possa rappresentare le istanze e tutto ciò che velocemente ci ha esposto oggi il sottosegretario L'Abbate sui tre temi che ho posto come criticità per sapere cosa ne pensasse il Governo. Oggi abbiamo in Aula un Governo che di fatto non c'è più.

venendo al tema specifico, voglio dire con concretezza che a noi di Fratelli d'Italia interessa che in materia di trattati - e, in questo caso, con questo trattato internazionale

al Parmesan - che non hanno nulla a che vedere con i nostri, ma che in qualche modo ingannano i consumatori e minacciano il sistema economico e produttivo del sistema Paese. Ci battiamo da molti anni affinché i prodotti che finiscano sulle nostre tavole abbiano un'etichettatura e anche una tracciabilità, come ha detto anche lei, che consenta di risalire alle origini e agli ingredienti prima che quel prodotto possa diventare un alimento. Noi, come Gruppo parlamentare e come partito con il nostro *leader*, Giorgia Meloni, manterremo sempre alta l'attenzione

Signor Presidente, la senatrice Binetti, unitamente ad altri colleghi, chiede quali iniziative si intendano intraprendere al fine di salvaguardare le attività e le funzioni dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e sostenere il turismo tra le categorie più svantaggiate, in particolare tra i giovani. In base al suo statuto l'AIG (Associazione italiana alberghi per la gioventù), costituita con atto del 19 dicembre 1945, è un ente morale assistenziale a carattere nazionale senza fini di lucro. L'associazione ha per scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile attraverso la realizzazione e la gestione degli ostelli per la gioventù e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire il miglioramento morale, culturale e fisico della gioventù mediante la pratica del turismo, considerato un mezzo insostituibile per la promozione sociale dei giovani e per favorirne la reciproca conoscenza. A livello internazionale l'AIG è membro e unico rappresentante per l'Italia

fu approvato e poi stralciato l'emendamento 15.0.13, che prevedeva la soppressione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e conseguentemente costituiva l'ente pubblico non economico denominato Ente italiano alberghi per la gioventù (EIG), sottoposto alla vigilanza del Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione delle competenze esercitate in materia di politiche per la gioventù.

in capo all'AIG. Gli oneri che lo Stato avrebbe sostenuto a decorrere dal 2020 sarebbero stati pari a 1,7 milioni di euro all'anno. Il Governo, oggi come un anno fa, è disponibile a valutare positivamente un'analoga proposta normativa per affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge.

dire al rappresentante del Governo che io non ho ben compreso quali siano le azioni concrete che possono essere messe in campo per salvaguardare questo patrimonio, che non è solo un patrimonio del nostro Paese, ma è un valore per tanti giovani e per le persone meno abbienti, che hanno trovato in questi spazi e in questi luoghi dei punti di riferimento importanti per l'attività turistica. Non comprendo inoltre come si possano salvaguardare le famiglie (stiamo parlando di circa 200 lavoratori e delle relative famiglie), che rischiano per la situazione di crisi in cui versa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, la quale potrebbe terminare la propria gloriosa esperienza.

proposti dal Governo al Parlamento, ai quali sono stati agganciati emendamenti che tentavano di risolvere questa situazione. Siamo a gennaio 2021 e ancora non c'è

identificare lo strumento idoneo per dare attuazione a questa richiesta che in maniera trasversale giunge dal Parlamento. Chiedo uno sforzo aggiuntivo, che sia veramente risolutivo. Con tutto il rispetto e ringraziando il Sottosegretario L'Abbate per la sua presenza in quest'Aula e per l'amabilità con cui ha risposto, sia pure in modo non soddisfacente, faccio presente che personalmente mi sarei aspettata la presenza del ministro Franceschini, cioè del Ministro che ha una delega al turismo, o del Ministro che in qualche modo ha una delega alla gioventù. Per carità, l'agricoltura va sempre bene, ma non è certamente il cuore del problema. Questo già dimostra lo scarso interesse per la specificità del quesito. Quello che stiamo vivendo è uno dei momenti di più drammatica emergenza economico-sanitaria che il Paese abbia mai attraversato - si dice - dalla

dei ministri rappresenta un'ulteriore limitazione a quelle che potremmo chiamare le libertà individuali - stiamo privando i nostri giovani della scuola in presenza, delle esperienze comunque culturali, anche di approfondimento, quelle legate alla vita universitaria e ai tirocini, e in questo caso anche di quella capacità di allargamento degli orizzonti.

economico-organizzativo i giovane nei loro spostamenti, poi a quella attuale di enti culturali. Stiamo, quindi, ancora una volta, considerando il mondo dei giovani nella peggiore delle modalità possibili, cioè non considerandolo. Chiaramente la risposta e

al filo, che potremmo chiamare in questo momento il famoso filo della cassa integrata e che sarà sottoposto comunque alla tagliola del 30 marzo, quando verrà meno il divieto dei licenziamenti.

di un Paese che non considera il turismo veramente il suo oro nero. L'esempio del turismo come oro nero del Paese è un esempio che fece il ministro Franceschini, Ministro da ben due legislature. Adesso non sappiamo cosa succederà nel prossimo Governo:

ma noi sappiamo che questa sorta di oro nero, che è il turismo italiano, non è mai riuscito ad essere preso in giusta considerazione come la ricchezza propria del Paese, una ricchezza economica, una ricchezza enogastronomica - e questo sicuramente riguarda anche le sue competenze

culturale, economico, sociale e organizzativo, e significa cecità nei confronti dei diritti delle nuove generazioni. Altro che il *recovery plan* come diritto della *next generation*!

di sospendere i nostri lavori, perché, anche raccogliendo le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto poco fa, mi sembra che siamo di fronte a una situazione paradossale. Siamo infatti qui per ascoltare le risposte di un Governo, che in sostanza non c'è più, come dimostra il fatto che abbiamo un Sottosegretario, che sta rispondendo a nome del Ministro delle politiche

sospendere i nostri lavori, in attesa che la crisi si chiarisca, in modo che il Parlamento abbia come interlocutore un Governo vero e non soltanto l'ologramma di un Governo che non esiste più. Balboni, capisco le ragioni della sua richiesta e personalmente le darei anche ragione, ma credo che una decisione del genere competa al Presidente

Signor Presidente, onorevoli senatori, la senatrice Corrado, unitamente ad altri colleghi senatori, chiede notizie sulla demolizione di parte delle fabbriche del villaggio agricolo cosiddetto Zaccarino e sullo stato di conservazione della chiesa di San Francesco d'Assisi, in agro di Giugliano, in provincia di Napoli. A tal proposito, occorre precisare che il territorio di Giugliano non è tutelato dal punto di vista paesaggistico e che la masseria in questione non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela, neanche dal punto di vista archeologico. In assenza di provvedimenti di tutela, la Soprintendenza non è stata coinvolta nel procedimento autorizzativo dei lavori in corso e ha appreso dell'avvenuta demolizione, confermata dal sopralluogo eseguito in data 13 luglio 2020, solo a seguito delle notizie comparse sui quotidiani. Sempre da una ricerca d'archivio, è emerso che nel 2018 è stata avanzata, da parte di privati, una richiesta di certificazione vincolistica, fondata sull'individuazione del bene unicamente tramite dati catastali. Tale certificazione è stata poi rilasciata con esito negativo. A seguito del sopralluogo, effettuato il 13 luglio scorso da funzionari della Soprintendenza, è emersa l'opportunità di sottoporre a provvedimento di tutela la piccola chiesa di San Francesco d'Assisi, posta nelle immediate vicinanze della masseria, lungo via Grotta dell'Olmo, e forse parte del medesimo complesso. In merito al quesito posto dall'interrogante sulla proposta di collaborazione tra Soprintendenza e Comune, si informa che la Soprintendenza, con nota del 15 luglio 2020, ha invitato il Comune di Giugliano a voler promuovere congiuntamente il censimento degli immobili di pregio sussistenti nel territorio comunale ed ha richiesto, nell'ambito di una auspicabile collaborazione istituzionale, la tempestiva informazione sulle attività edilizie in corso, inerenti a beni immobili di privati non sottoposti a provvedimenti di tutela, aventi oltre settanta anni di età, al fine di poter svolgere una preventiva attività di verifica sull'eventuale sussistenza di interesse architettonico e storico-artistico.

Intanto noto lacune persino nella ricostruzione dei fatti, dal momento che la demolizione di cui parliamo risale al 9 luglio scorso. Il giorno stesso, l'ottima giornalista Claudia Procentese pubblicò un *post* sulla sua pagina Facebook, mediante il quale, con immagini assolutamente parlanti, la comunità nazionale è venuta a conoscenza di questa demolizione, realizzata in poche ore il giorno stesso, quindi sempre il 9 luglio scorso, tant'è che poi, come diceva il Sottosegretario, il sopralluogo della Soprintendenza per l'area metropolitana di Napoli è del 13 luglio. In poche ore, il complesso edilizio - che si doveva al barone Giovanni Battista Orineti,

dell'edificio precedente, il quale era però una masseria settecentesca, realizzando 48 appartamenti e una grande piscina condominiale con un piano seminterrato per i *garage.* Questo significa che è stata applicata la legge regionale n. 19 del 2009, il cosiddetto piano casa, che in Campania consente ricostruzioni anche con aumento di cubatura,

che sicuramente aveva un valore identitario per la popolazione e che in verità finora era sfuggito alle mire dei palazzinari solo per la vicinanza ad alcune discariche, in particolare quella di Settecainati. Tuttavia, prima la Soprintendenza o il Comune (un ente territoriale) avrebbero dovuto avviare il procedimento di verifica dell'interesse culturale. Non è stato fatto né richiesto. La Soprintendenza afferma di aver avuto contezza di quanto accadeva nel momento in cui la demolizione è avvenuta, tuttavia ammette che mesi prima, vale a dire a gennaio del 2019, in base a una richiesta dell'ottobre precedente, aveva risposto a una domanda sulla

al Comune di Giugliano per sapere se avesse dato o stesse per dare il permesso di demolizione di un immobile storico, sul quale non c'era un vincolo esplicito, ma che certamente, essendo settecentesco, aveva superato i settant'anni, quindi era tutelato *ex lege*. C'è stata quindi una una complicità involontaria nel girare lo sguardo dall'altra parte e si è perso un pezzo importante della storia del territorio. Desidero dare un senso a questo sacrificio del casale Orineti di Giugliano, come ho fatto, del resto, con la collega Mariolina Castellone, andando sul posto il 18 luglio

Occorre una strategia nazionale a tutela del patrimonio edilizio rurale storico. Non parlo dei centri storici e della proposta di tutela dell'Associazione Bianchi Bandinelli, perché ci vorrebbe molto più tempo; tuttavia, in tutto il Paese siamo veramente in una condizione di pericolo altissimo, ogni giorno di perdere tutto il costruito rinascimentale e moderno moderno (migliaia di edifici, che sono la storia nostra e del nostro territorio) e di perdere il contesto in cui è inserito. È un'emergenza del Paese, che passa sotto silenzio anche a causa della strategia

alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, è tutt'altro ed è inscindibile dalla valorizzazione. Spero pertanto che questo sacrificio della masseria di Giuliano non vada completamente perduto e ci possa essere un ripensamento delle politiche del Ministero per i beni e le attività culturali

forze politiche che sostengono il Governo abbia deciso di ritirare due suoi componenti dal Consiglio dei Ministri evidentemente ci dice che, per l'appunto, la crisi si è aperta. Attendiamo e ci aspettiamo che presto il Presidente del Consiglio venga per formalizzare quanto è nelle cose, ovvero si rechi al Quirinale per trarre le conseguenze di quanto avvenuto. Di certo, è dignitoso che il Senato sia informato e partecipe della vicenda e che la questione non resti in palazzi estranei a quelli dove, invece, c'è la rappresentanza del popolo italiano, sulla base di quanto indicato Signor Presidente, sinceramente speravo che accogliesse la mia richiesta di poco fa.

Non ho bisogno di ricordare a lei e a tutti i colleghi la situazione drammatica, dal punto di vista sanitario ed economico, che l'intero Paese sta vivendo. Non possiamo rimanere un minuto di più in questa situazione di grave

finestra") Colleghi, comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di non svolgere le interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento,

Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il medesimo decreto, il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il predetto Dicastero. Il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta, ha altresì accettato le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio e dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che martedì 19 gennaio, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni al Senato sulla situazione politica in atto.

Seguiranno le dichiarazioni di voto su eventuali strumenti di indirizzo presentati. L'organizzazione dei lavori dovrà tenere conto dei tempi di sanificazione dell'Aula.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

in Aula al Senato a riferire con comunicazioni su quanto accaduto e sulla crisi politica in atto solo nella giornata di martedì prossimo. Partendo dalle parole del Presidente della Repubblica, in cui

Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì: passano sei giorni! *(Commenti)*. È davvero incredibile. Vista la situazione drammatica in cui versa il nostro Paese,

ha una maggioranza, oppure, se non ce l'ha, a rassegnare le dimissioni, in modo tale che il Presidente della Repubblica possa intraprendere il giro di consultazioni e velocizzare le procedure, per dare eventualmente un nuovo Governo al Paese. Questo è il problema vero ed è lo scandalo vero. Tra l'altro, quello che poi si è consumato nella nella Conferenza dei Capigruppo, sia di questa mattina che di questa sera, ha un po' del grottesco, perché nella Conferenza dei Capigruppo di questa mattina, la maggioranza mattina, la maggioranza - sempre che ci sia ancora e che sia tale: questo è tutto da valutare e lo vedremo - addirittura immaginava

che aveva la maggioranza, che non si capisce ancora se è tale, facendo proprio finta di nulla, come se nulla fosse successo. Abbiamo addirittura

quasi nero su bianco questo accordo stabilito da tutti, c'è stato un dietrofront: Conte non dà più la disponibilità per lunedì perché, se si finisce all'una di notte, purtroppo è troppo tardi e forse non si riesce a portare qualcuno a votare *(Applausi)*.

È chiaro che avete bisogno di giorni, che vi siete presi dei giorni per andare a cercare i cosiddetti responsabili. Volete l'orario giusto perché per qualcuno magari magari probabilmente all'una di notte è troppo tardi e, quindi, bisogna chiamarlo prima. Questo sarebbe il Governo che può dare un futuro al Paese e soprattutto il Governo del rilancio dell'Italia? Tanti auguri!

Signor Presidente, io la ringrazio. Devo dire che il collega Romeo mi ha anticipato con una serie di considerazioni che sono state per noi uno *shock* continuo. Colleghi, ho sentito dire oggi ho sentito dire oggi che il presidente Conte non può presentarsi nello stesso giorno in quest'Aula del Senato e alla Camera perché ciò potrebbe pregiudicare i diritti dei senatori anziani. *(Applausi)*. Noi ci siamo commossi di fronte a questa sensibilità che avete ripetutamente dimostrato quando avete forzato il calendario dei lavori in maniera vergognosa, facendo votare anche ai senatori anziani - poveretti fiducie ad ogni ora del giorno e della notte *(Applausi)*. Eppure in questo momento, per la vostra paura che a questo Governo raccogliticcio manchi qualche senatore, magari qualche senatore a vita un po' *agé,* avete il coraggio di menzionare la debolezza, la vulnerabilità, la fragilità dei senatori anziani *(Applausi)*. Signor Presidente, lei - pur se imparziale ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Tra l'altro, vorrei fare un ringraziamento personale al presidente Conte che, quando è stato interpellato, aveva manifestato la sua disponibilità. Aveva infatti comunicazioni lunedì mattina alla Camera e coerentemente, per equilibrio e *par condicio,* lunedì pomeriggio al Senato. Questa ci sembra la cosa giusta, salvo che qualcuno di voi non abbia retropensieri, preoccupazioni, angosce, esigenza di ramazzare costruttori all'interno di quest'Aula fino all'ultimo secondo *(Applausi)*. È una cosa di cui forse il presidente Conte non era stato messo a conoscenza, ma la sua maggioranza, a distanza di una ventina di minuti, ha pensato bene di rettificare la sua disponibilità; la disponibilità data dal presidente Conte che, ogni giorno, dice di preoccuparsi profondamente per i problemi del Paese e addirittura fa dei video di andare a prendere il caffè e manifesta tutta la sua empatia, partecipazione e vicinanza agli italiani e rimanda in maniera vergognosa

è. Sappiamo che sono stati ritirati dei Ministri, ma non sappiamo se è stata ritirata la fiducia. È questo il modo in cui voi servite i vostri rappresentati? È questo il modo in cui voi servite quegli italiani che dite stanno soffrendo? È questo il modo in cui voi seguite la pandemia e la crisi? se questa è l'alba di un nuovo giorno, noi ci auguriamo veramente che questo giorno non venga mai e continueremo a lavorare esattamente come voi perché Governi raccogliticci, che faranno solo il male del Paese, non nascano mai con i peggiori presupposti. Aggiungo ancora un particolare non irrilevante. Colleghi, vi stiamo chiedendo da due mesi di fare presto. Fate presto! *(Applausi)*. Colleghi del MoVimento 5 Stelle, voi che volevate aprire quest'Aula come una scatoletta di tonno,

Abbiamo anche contingentato i tempi per far sì che tutto questo si svolgesse in un solo giorno. Poi, all'improvviso, questo sistema è stato rovesciato si è tornati a uno schema che - a nostro avviso - è inaccettabile, ossia due giorni divisi: lunedì alla Camera e martedì al Senato. Questo vuol dire che, dall'inizio di questa crisi, rispetto alla quale si fa finta di niente, sarà passata

che ha chiesto che questa crisi abbia tempi brevissimi, e di fronte alle emergenze sanitarie ed economiche del Paese, che non può aspettare il pantano della politica (quindi, tempi non brevi, ma brevissimi),

Tutta l'opposizione ha dato disponibilità per le giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì. Avete traccheggiato con ogni scusa, anche la più bassa e ridicola, per arrivare a martedì. Avete bisogno del sabato e della domenica non per riposare, ma per cercare di puntellare una maggioranza che non c'è più, andando a prendere di qua e di là qualche anziano che sopravvive alle due di notte o qualche altro definito impropriamente responsabile, per capire se avete o meno dei numeri risicati. *(Applausi)*. Voglio dirvi una cosa. Conte avrebbe dovuto dimettersi e sarebbe dovuto venire oggi a dire che cosa sta succedendo, che cosa si intende fare e procedere subito alla conta.

maggioranza, questa sarà tre volte più debole di quella che avete avuto fin qui e con la quale avete rovinato il Paese.

Signor Presidente, una settimana fa, il 7 gennaio, su «Il Giorno», nelle pagine milanesi, compariva un articolo che, per la prima volta, dava conto dello stato dell'arte della trattativa fra lo Stato e gli eredi di Umberto Eco.

da altri interventi sulla stampa - sembrano arrivare in porto. Eppure, diversamente da quanto era dato sapere fino a qualche tempo fa, e cioè che il Ministero per i beni e le attività culturali stava trattando con la famiglia, dopo avere dichiarato l'interesse storico particolarmente rilevante del compendio costituito dalla biblioteca e dall'archivio di Umberto Eco, oggi si apprende che la biblioteca, relativamente alla parte dei testi antichi e rari, sarà effettivamente acquistata dallo Stato e sarà conservata nella biblioteca nazionale Braidense di Milano e gestita, appunto, dal Ministero. Al contrario, oltre 35.000 volumi - sono la parte più recente della biblioteca stessa - e le carte, quindi l'archivio del professore, saranno donati dalla famiglia allo Stato,

per raccogliere questa parte della documentazione e dei libri. Mi chiedo come sia possibile che il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha emesso un provvedimento di tutela - rispetto al quale la famiglia Eco ha fatto un ricorso al TAR, e sul quale non si è ancora deciso - possa permettere lo svilimento di questa propria iniziativa di tutela,

pur contenendo anche i libri una serie di note manoscritte e di appunti dello stesso Eco: a me sembra una cosa molto poco giustificata, tanto più che - ripeto - un provvedimento di vincolo era già stato emesso e adesso sembrerebbe che, pur restando in vigore il vincolo, il Ministero permetta - a quanto sembra, sulla base dei desideri dei familiari - uno smembramento che non ha senso. *(Applausi)*.

nella quale, dal 2011, ha ricoperto per tre volte l'incarico di amministratore delegato. Secondo lo statuto della Consap, gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea. Dunque, Masi, non potendo ricoprire per una quarta volta il ruolo di amministratore delegato, ha ottenuto la presidenza, mentre la poltrona di amministratore delegato è andata a Vincenzo Federico Sanasi D'Arpe. Sempre lo statuto della Consap

ovvero gli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto, ossia le banche fallite. Masi è anche presidente di Banca Igea, un'altra banca la cui compagine azionaria ha salvato la Banca del Fucino,

che era SGA ex Banco di Napoli ed è diventata AMCO, società partecipata dal MEF. Come direttore generale Rai, Masi è stato condannato in via definitiva per danno erariale proprio nei confronti della TV pubblica e ha dovuto risarcire l'azienda per 100.000 euro. Da direttore generale favorì l'esodo dell'ex direttore del telegiornale Angela Buttiglione e dell'ex direttore Rai Marcello del Bosco, facendo sborsare alla Rai 680.000 euro; cifra che la Corte dei conti ha giudicato danno erariale con sentenza confermata dalla Cassazione il 16 ottobre 2018. signor Presidente, secondo noi è inconcepibile che siano sempre i soliti mandarini a essere rinnovati quasi in eterno. se l'incarico di presidente della Consap ricoperto da Mauro Masi sia compatibile con quello di presidente di Banca Igea, considerando che la concessionaria di servizi assicurativi pubblici gestisce anche il FIR, il fondo per indennizzare i risparmiatori. Quali iniziative bisogna svolgere? Questo Paese non cambierà fino a quando i soliti mandarini di Palazzo continueranno a infestare gli enti pubblici. *(Applausi)*.

delle sigle sindacali di aziende aeroportuali come Alitalia e delle *handling* Aviation Services e Aviapartner che proprio ieri mi hanno denunciato che dal 27 gennaio

quali vedremo i nostri concittadini, i lavoratori del sistema aeroportuale, non percepire lo stipendio. Intervengo quindi in fine seduta per sensibilizzare soprattutto il Ministro del lavoro affinché si faccia carico presso l'INPS, visto che spesso e volentieri gli intoppi che produce la nuova dirigenza INPS creano disagi ai cittadini. Dal 27 gennaio prossimo

il fatto che dal 27 gennaio i lavoratori delle aziende Aviation Services, Aviapartner e Alitalia - ripeto - non percepiranno lo stipendio e questo problema è spalmato su tutto il territorio, da Napoli fino a Milano, passando per l'aeroporto internazionale di Fiumicino. Questo è un appello accorato alla serietà